comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata lunedì 28 dicembre, alle ore 16. Il Senato tornerà quindi a riunirsi lunedì 28 dicembre, alle ore 17, con all’ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente».

e la vicinanza alle famiglie e alle comunità colpite. Il Governo è in contatto col prefetto e con tutte le autorità locali presenti. La ringrazio di questo spazio.

Migliaia di aziende in settori innovativi legati alla canapa industriale vedevano nelle iniziative di questi giorni un timido passo avanti che invece non c’è stato. La bocciatura del settore della canapa industriale è una scelta ignorante. Parliamo di una filiera composta da 12.000 operatori sul territorio che hanno scelto di dedicarsi a una pianta versatile senza efficacia drogante; una filiera che aspettava solo di essere regolamentata. In periodo di autarchia il fascismo obbligò alla coltivazione di canapa industriale i cittadini, perché coltura povera, ma altamente versatile. Per una Nazione come l’Italia la canapa è stata un fattore determinante del rilancio post-Prima guerra mondiale. Oggi si assiste a uno scenario assurdo della destra, che sembra non ricordare più cosa ha significato la canapa per l’Italia e gli italiani. Dall’altro lato, è stato approvato un emendamento a favore della cannabis terapeutica, con uno stanziamento di circa 4 milioni di euro per aumentare l’importazione e la produzione nazionale. Ciò non è però sufficiente. A fronte dei milioni di euro già spesi per la produzione italiana, non si è mai raggiunto il quantitativo di cannabis stabilito per lo stabilimento di Firenze quando, con le stesse risorse, si sarebbero potute generare 10 volte le stime di produzione che però non si sono mai concretizzate. A distanza di cinque anni dall’avvio del progetto pilota non sono mai state riviste, nonostante i solleciti dell’associazione di malati e familiari, le stime della domanda di cannabis medica in Italia; non sono stati effettuati controlli su Firenze; non sono stati avviati nuovi progetti e nuove autorizzazioni. Questo Parlamento non deve piegarsi a logiche di ignoranza e pregiudizio. La cannabis è un tema per chi ha il coraggio di parlare della storia dell’Italia e di valorizzare un’eccellenza - la pianta della cannabis, appunto che nel nostro Paese ha avuto un ruolo millenario.

intervenire su un tema da sempre al centro dei dibattiti politici e su cui molto è stato fatto, anche se in maniera ancora insufficiente.

cittadini: persone e famiglie che, a causa del loro sovraindebitamento, si vedranno portar via la loro unica casa o beni mobili e immobili strumentali all’esercizio della propria impresa e professione. Su questo, signor Presidente, bisogna intervenire con molto più coraggio. Certo, è vero, ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte economiche e a pagarne le conseguenze non può e non deve essere il creditore, ma, al contempo, un Governo non può lasciare i propri cittadini in difficoltà, in balia di banche, istituti di credito intermediari finanziari o, peggio ancora, organizzazioni criminali che di questo fenomeno hanno fatto un vero e proprio business spietato. Oggi dobbiamo avere il coraggio di affermare che su questo fenomeno c’è un vero e proprio mercimonio legalizzato, dove sono gli stessi magistrati - per fortuna pochi, pochissimi - i funzionari di cancelleria, i consulenti tecnici, gli avvocati o i notai delegati a trarne un illecito vantaggio, speculando sulle famiglie in difficoltà che non riescono a onorare le rate dei mutui accesi presso le banche, oppure sull’incremento inarrestabile di fallimenti di piccole e medie aziende, spesso abilitati proprio dai tribunali. Sono fatti di cronaca, signor Presidente.

tutelando sempre il creditore. Non possiamo creare delle immunità di fatto verso chi ha contratto degli impegni. Non possiamo assolutamente creare delle distorsioni verso il sistema delle tutele dei creditori.

che si ridia dignità al Parlamento, iniziando proprio da chi questo Natale lo vivrà con l’angoscia di non poter garantire alla propria famiglia di continuare a vivere nella propria casa. (Applausi).